Il Ministero degli affari esteri, e il ministro Franco Frattini in prima persona, seguono con la massima attenzione la vicenda di Daniele Franceschi, deceduto nel penitenziario di Grasse, in Francia, lo scorso 25 agosto. Il ministro Frattini ha ricevuto in due occasioni, pochi giorni dopo l'episodio e il 20 ottobre scorso, la madre, signora Antignano, e ha ribadito l'impegno affinché venga fatta piena luce sulla morte di Daniele. «Vogliamo ascoltare tutta la verità dal giudice istruttore» ha dichiarato il Ministro, auspicando che la giustizia francese assicuri un chiarimento definitivo su questo caso così doloroso. Da parte sua, il Ministro della giustizia francese ha fatto sapere di aver impartito puntuali istruzioni affinché la questione venga trattata con la più grande trasparenza. Fin dall'inizio, la Farnesina si è adoperata per assistere la famiglia e sensibilizzare le autorità francesi. Appreso del decesso del connazionale, detenuto in attesa di giudizio per il presunto uso di carta di credito falsa presso un casinò della Costa azzurra, il console generale a Nizza ha subito informato i familiari di Daniele a Viareggio. Egli ha chiesto al procuratore di Grasse di essere aggiornato sulle indagini e sul procedimento avviato per accertare le cause del decesso. La famiglia Franceschi si è costituita parte civile, avvalendosi di un avvocato locale suggerito dallo stesso consolato generale. Grazie all'intervento del console generale, i familiari hanno potuto vedere il corpo di Daniele prima degli esami disposti dalle autorità locali. L'ambasciata a Parigi e il consolato generale a Nizza erano intervenuti affinché un medico di fiducia della famiglia fosse presente all'autopsia, istanza purtroppo rigettata dal procuratore di Grasse. Nel successivo referto è stata affermata l'assenza di tracce di violenza fisica, segnalando che gli organi interni erano ancora sottoposti ad esame. La madre di Daniele ha chiesto il rimpatrio della salma per procedere ad un esame autoptico in Italia, richiesta ribadita anche a fronte della segnalazione delle autorità francesi che gli organi interni sarebbero stati resi disponibili solo a dicembre. Lo stesso ministro Frattini, in una lettera al suo omologo francese Bernard Kouchner, ha sottolineato l'esigenza che il corpo venisse mantenuto in condizioni tali da consentire un nuovo esame in Italia. Il ministro Kouchner ha risposto di aver immediatamente interessato il Ministro della giustizia francese e ha assicurato di aver rimarcato la necessità di restituire la salma in maniera consona. Avendo però appreso, nella fase di definizione del volo di rimpatrio, che la salma, scongelata per la prima autopsia, era stata conservata ad una temperatura superiore a zero gradi (condizione, a detta dello specialista patologo italiano contattato al riguardo, non idonea ad assicurare la piena efficacia del secondo esame), il consolato generale a Nizza è subito intervenuto sulle autorità francesi per ottenere delucidazioni in merito. I legali della famiglia, in occasione dell'audizione della signora Antignano al tribunale di Grasse del 3 novembre, hanno ribadito che le spoglie avrebbero dovuto essere conservate in stato di congelazione. Il corpo di Daniele è tornato in patria, grazie all'intervento del nostro Ministro degli esteri, con un volo militare ed è stato finalmente sottoposto ad autopsia in Italia. Questa ha potuto constatare l'assenza di lesioni traumatiche, senza però poter fornire, data l'assenza degli organi interni, un'indicazione definitiva sulle cause del decesso. Su istruzione del ministro Frattini, la nostra ambasciata a Parigi ha ribadito ai Ministeri francesi degli esteri e della giustizia l'esigenza che gli organi interni, *in primis* il cuore, siano mantenuti in condizioni tali da permettere un ulteriore esame in Italia e siano restituiti alla famiglia il più celermente possibile. Medesima richiesta è stata ribadita dal nostro consolato generale a Nizza al procuratore di Grasse. Il Ministro degli esteri francese ha scritto al ministro Frattini indicando che gli esami anatomo-patologici e tossicologici connessi all'inchiesta non consentiranno di restituire gli organi prima di metà dicembre. Dai Ministeri francesi della giustizia e degli esteri si è però assicurato l'impegno a far sì che ciò avvenga in condizioni tali da permettere nuove indagini. Per quanto riguarda la restituzione degli effetti personali, in particolare del diario di Daniele, il console generale a Nizza è intervenuto sul procuratore di Grasse affinché l'istanza della famiglia venga accolta quanto prima. Il giudice istruttore francese ha ordinato alla polizia giudiziaria di cercare il diario e altri scritti di Daniele che possano contribuire allo sviluppo delle indagini. Il console generale ha inoltre chiesto chiarimenti circa il fermo della signora Antignano, avvenuto il 13 ottobre mentre manifestava di fronte al carcere di Grasse. Il console generale era tempestivamente intervenuto per ottenere il rilascio della mamma di Daniele, che ha poi lamentato maltrattamenti della polizia. Il ministro Frattini ha personalmente assicurato ai familiari che la Farnesina continuerà ad essere al loro fianco affinché sia accertata la verità.

che continuerà ad essere attentamente monitorata dal Governo italiano. Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri, onorevole Stefania Craxi, per essere venuta in Aula a rispondere alla mia interrogazione. Apprezzo molto che il ministro Frattini abbia manifestato l'intenzione di seguire di persona e con la massima attenzione la vicenda di Daniele Franceschi. Purtroppo - e credo di interpretare il pensiero della madre, alla quale sono vicina con tutto il mio affetto - le risposte che fino ad oggi ci sono state date non possono essere ritenute soddisfacenti. Mentre apprezziamo l'operato del console generale a Nizza, che ha immediatamente avvisato la famiglia e che ha molto agevolato la madre nel tentativo di vedere il corpo prima degli esami disposti d'ufficio dalle autorità carcerarie, non possiamo non rilevare che l'intervento del Governo italiano non è stato sufficientemente incisivo, in primo luogo, verso le autorità francesi, che non hanno consentito che un medico di fiducia della famiglia fosse presente all'autopsia (diniego opposto, così si dice, in base alla normativa locale); in secondo luogo, verso il Ministro della giustizia francese, che non si è attivato finché la salma fosse conservata in maniera consona, in condizioni tali cioè da consentire il nuovo esame autoptico in Italia, autorizzato dalla procura di Lucca; in terzo luogo, verso polizia di Grasse, per il modo indegno con cui è stata fermata, arrestata e maltrattata la madre di Daniele il 13 ottobre mentre manifestava di fronte al carcere di Grasse (un ringraziamento va comunque al console generale per essere intervenuto immediatamente ottenendo il rilascio della signora, che ne è uscita con le costole rotte, e non metaforicamente); luogo, verso la magistratura francese che non ha ancora restituito, come l'onorevole Craxi ha detto, gli organi mancanti prelevati per esami tossicologici che risultano tuttora in corso, a causa di una lentezza imperdonabile e ingiustificabile; verso le autorità carcerarie di Grasse che, oltre a non aver prestato le giuste cure e il necessario soccorso al ragazzo - ci fa molto pensare anche il sequestro del defibrillatore, che ora sembra essersi inceppato non hanno ancora restituito alla madre gli effetti personali e, soprattutto, il diario, che anche l'onorevole Craxi citava, sul quale Daniele scriveva ed annotava tutto, quasi in modo maniacale, delle sue giornate, e che è sparito. Ci viene da dubitare e da domandarci: forse è sparito perché conteneva tutte le risposte? Detto questo, vigileremo affinché queste e le altre interrogazioni non vengano dimenticate, ma soprattutto affinché sia fatta piena luce sulla morte di un ragazzo che era in carcere dal febbraio 2010 con l'accusa di falsificazione di carte di credito in un casinò e che non è mai stato processato. E vigileremo anche affinché gli organi siano restituiti al più presto all'Italia ed in condizioni tali da permettere gli esami autoptici, perché quello che noi temiamo fortemente è che anche questi organi possano giungere in condizioni disastrose, come è giunta la salma. Invitiamo dunque, di nuovo e fortemente, il Governo ad intervenire con fermezza sulle autorità competenti francesi perché un fatto così grave, tra l'altro avvenuto in un carcere, quello di Grasse, dove non è la prima volta che vengono svolte indagini per fatti simili, non abbia più ripetersi. A questo proposito, affinché Daniele non sia morto invano, ho chiesto e ottenuto dalla Commissione per i diritti umani di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dei nostri connazionali detenuti nelle carceri all'estero: cominciano ad essere davvero troppi i casi e le segnalazioni di detenuti

Signor Presidente, lo Studio per il sistema aeroportuale italiano costituisce la conclusione dell'indagine tecnica basata sull'analisi dello stato attuale degli scali nazionali al fine di offrire delle ipotesi di lavoro non solo per le future scelte di politica di trasporto aereo ma anche per le altre modalità di trasporto. Sarà pertanto a tale livello di sistema che potranno essere definite le scelte strategiche. La finalità dello studio è stata, tra l'altro, quella di offrire uno strumento valido ed aggiornato relativo al sistema aeroportuale nazionale per gli opportuni confronti con le realtà degli altri Paesi europei. l'obiettivo dello studio è stato quello di valutare, in maniera adeguata ed interconnessa con gli altri sistemi di trasporto, i nodi fondamentali del trasporto aereo nazionale, cercando di valorizzare la funzione dei singoli scali aeroportuali nell'ottica di un sistema di rete, coerentemente con la situazione storica, attuale e ragionevolmente prevedibile, ed evidenziando le criticità del sistema del trasporto nazionale nel suo complesso in relazione all'ottimale sviluppo degli aeroporti stessi, con l'offerta di uno strumento di supporto alla pianificazione, non solo per il settore aereo, ma anche per le altre modalità di trasporto. In conclusione, si intende assicurare che ogni ventilata ipotesi riguardante chiusure o ridimensionamenti di scali nazionali - tra cui quello di Perugia - non è oggetto dello studio in questione, in quanto solo concrete strategie successive potranno definire la vocazione e la missione di ciascuna realtà aeroportuale in un'ottica di valorizzazione delle infrastrutture esistenti.

per la regione Umbria e fondamentalmente per l'intero Centro-Italia, in quanto può costituire un punto strategico di collegamento, e ha un'importanza fondamentale anche per lo sviluppo economico della Regione

conto del criterio base sul quale si è fondato lo studio di Nomisma, che guarda al numero di passeggeri in transito piuttosto che all'importanza strategica di uno scalo aeroportuale rispetto al territorio di riferimento, soprattutto

Le istituzioni locali, la Regione *in primis*, stanno scommettendo sul futuro di questo aeroporto, con somme importanti per investimenti volti al completamento dell'area aeroportuale, con servizi ulteriori. I lavori sono in corso per rendere l'aeroporto più moderno e adeguato a ricevere fino a 500.000 passeggeri in transito. D'altra parte il Governo si è impegnato a finanziare questi investimenti con l'accordo di programma sottoscritto

Signor Presidente, come correttamente riferito dagli interroganti, senatori Bodega, Mazzatorta, Mura e Valli, a partire dal 29 aprile 2010 è entrato in vigore il regolamento n. 300 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (che abroga il regolamento della Comunità europea n. 2320 del 2002) e con esso anche alcuni regolamenti attuativi, fra i quali vi è il regolamento dell'Unione europea n. 185 del 2010 . Tale ultimo regolamento, nel disporre un elenco di articoli proibiti per il bagaglio da stiva (tra i quali vi sono anche le munizioni), prevede la possibilità di derogare a tale divieto sulla base di due condizioni: l'autorità competente deve basarsi su norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione; questione; devono essere ottemperate le norme di sicurezza vigenti. A tale riguardo, si evidenzia che in data 29 aprile ultimo scorso, quindi contestualmente all'entrata in vigore del regolamento n. 300 del 2008 e dei regolamenti collegati, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha emanato una direttiva che contiene le relative disposizioni attuative. Tale direttiva include, al paragrafo 5.4, la deroga disciplinata dal punto 5.4.2 del regolamento dell'Unione europea n. 185 del 2010, esplicitando la possibilità di portare armi e munizioni nel proprio bagaglio di stiva purché vengano rispettate le procedure previste dalla legge n. 694 del 1974 e dal punto n. 10 - scheda 2 del piano nazionale di sicurezza. I passeggeri sono inoltre informati in merito agli articoli proibiti elencati nell'appendice 5-B del citato regolamento dell'Unione europea n. 185 del 2010 prima del completamento delle operazioni di registrazione. Alla luce di quanto riportato, si rappresenta che le problematiche poste dagli onorevoli interroganti in riferimento all'adozione di una normativa nazionale che consenta il trasporto aereo di munizioni nel bagaglio di stiva sono state già tenute in considerazione dall'ENAC, in qualità di autorità competente.

Noi della Lega Nord siamo i primi a tenere alla sicurezza dei voli aerei: bisogna mettere in atto tutte le procedure necessarie in momenti particolari come questi, in cui il terrorismo, tra l'altro, imperversa

quindi soddisfatti della risposta, che fa chiarezza al riguardo. Siamo consapevoli che, durante il corso di quest'anno, altre normative sono entrate in vigore, in modo particolare per quanto riguarda il rilascio dei permessi di porto d'armi e quant'altro.

in relazione agli impianti di manutenzione del materiale rotabile di Trenitalia, con particolare riferimento all'Officina di Melfi, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che Trenitalia sta attuando un programma di riorganizzazione del settore della manutenzione, finalizzato a: migliorare la disponibilità all'esercizio e l'affidabilità del materiale rotabile; incrementare i livelli di produzione e produttività del settore; settore; reingegnerizzare i processi produttivi attraverso la specializzazione e ripartizione delle attività manutentive in base alla tipologia di materiale rotabile per migliorare la qualità; qualità; ridurre i costi mediante la concentrazione degli impianti, in linea con gli standard europei. Tale programma prevede anche la razionalizzazione del reticolo manutentivo,

organizzativa e tecnologica. Nello specifico, le valutazioni sono state effettuate tenendo a riferimento le principali priorità alla base del piano di risanamento aziendale e cioè: concentrazione della manutenzione in poli specializzati; incremento della produttività di ciascun impianto e contenimento dell'incidenza dei costi fissi rispetto ai costi complessivi di produzione. In tale ambito si colloca la programmata chiusura dal 2011 dell'Officina di Melfi citata dall'interrogante, senatore Latronico, che presenta indici di produttività sensibilmente inferiori alla media nazionale e una elevata incidenza dei costi fissi. Per quanto concerne il personale impiegato nell'Officina, questo potrà essere utilizzato negli altri impianti manutentivi dei territori viciniori e, comunque, l'attuazione dei relativi provvedimenti sarà gestita attraverso gli strumenti previsti dall'attuale normativa contrattuale e i protocolli di relazioni industriali. Va, infine, sottolineato che, a seguito degli interventi di riorganizzazione in programma, il volume complessivo delle attività manutentive di Trenitalia, sia cicliche che correnti, rimarrà sostanzialmente costante.

Stiamo parlando di un'officina che ha un capitale di esperienze, di competenze e di specializzazione: sono 50 le unità lavorative impegnate nello stabilimento di Melfi,

il sistema della logistica, il tema dell'ammodernamento delle reti nel Mezzogiorno, il tema del miglioramento della qualità dei servizi che la la mobilità, in generale, e il sistema ferroviario, in particolare, devono garantire per il rilancio del Mezzogiorno.